iniziati con l'incendio del centro di prima accoglienza e soccorso, situato presso Contrada Imbriacola, a Lampedusa. Il Governo - come per analoga richiesta formulata dalla Camera dei deputati - ha dato prontamente la propria disponibilità a riferire sull'accaduto, con un'informativa che tiene conto degli elementi acquisiti per il tramite della prefettura di Agrigento e del Dipartimento della pubblica sicurezza. Desidero innanzitutto dare atto e ringraziare, anche in quest'Aula, il prefetto, il questore, i responsabili di tutte le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco per gli interventi attuati per fronteggiare l'evento, che sono stati pronti e immediati. Come ho già ieri riferito alla Camera, l'episodio al centro della ricostruzione odierna si colloca nella situazione di emergenza che, sin dai primi mesi di quest'anno, coinvolge in modo particolare l'isola di Lampedusa, proprio per la sua collocazione geografica di maggiore prossimità all'Africa. Prima di addentrarmi nella ricostruzione dei fatti, a nome del Governo voglio esprimere un sentimento di solidarietà nei confronti della popolazione di Lampedusa, per lo spirito di accoglienza di cui ha dato e sta dando prova, comportamento che non risulta affatto offuscato da qualche manifestazione di disagio e di insofferenza. Il 20 settembre scorso, alle ore 16,45 circa, presso il centro si sviluppava un incendio di notevoli dimensioni. Secondo quanto emerge dai primi accertamenti compiuti dalle forze di polizia e dai Vigili del fuoco, l'incendio sarebbe stato contestualmente appiccato sarebbe stato contestualmente appiccato da cittadini tunisini presso tre dei quattro padiglioni della struttura. Nella circostanza, circa 950 immigrati si sono allontanati, dirigendosi verso il centro abitato di Lampedusa. I Vigili del fuoco intervenivano immediatamente, sia con il personale del presidio, che dall'inizio dell'emergenza opera presso il centro, sia con il personale di rinforzo. Altrettanto tempestivo è stato l'intervento delle forze di polizia in servizio, finalizzato anche a rintracciare i tunisini e a raggrupparli presso alcuni siti, quali il campo sportivo e la zona antistante la caserma della Guardia di finanza. Per meglio fronteggiare l'emergenza, il prefetto di Agrigento convocava una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, con la partecipazione del comandante provinciale dei Vigili del fuoco e del comandante della Capitaneria di Porto Empedocle. Nella circostanza, veniva disposto un mirato rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio. Voglio ricordare che sono a disposizione della questura di Agrigento 460 unità, incrementate, nell'immediatezza dell'evento, di ulteriori cento. Concorrono, inoltre, ai servizi di vigilanza e controllo anche 150 militari delle Forze armate. I danni cagionati dall'incendio hanno reso inutilizzabili tre padiglioni della struttura. La maggior parte degli immigrati veniva rintracciata e ricondotta all'interno del centro, nell'unico padiglione utilizzabile, mentre la restante parte è stata sistemata presso il campo sportivo comunale. Sei immigrati, due appartenenti alla Polizia di Stato e un dipendente dell'ente gestore hanno dovuto fare ricorso alle cure per intossicazione da fumo. Nessun minore era presente nella struttura al momento dell'incendio. L'attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato ha consentito di risalire agli autori dell'incendio, individuandoli in quattro cittadini tunisini, sottoposti al fermo di polizia giudiziaria per i reati di incendio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I disordini sono proseguiti nella mattinata di mercoledì 21 settembre quando circa 400 tunisini si sono concentrati in prossimità di un distributore di benzina mentre alcuni lampedusani, che nella stessa mattinata si erano raggruppati davanti alla sede del Comune, raggiungevano la zona del distributore. Alcuni immigrati, impossessatisi di bombole di gas collocate all'esterno di un ristorante, minacciavano i lampedusani, creando un potenziale pericolo di esplosione per il distributore di benzina. I lampedusani lì accorsi iniziavano una sassaiola all'indirizzo dei tunisini. Sul posto intervenivano i vigili dei fuoco con i propri mezzi, mentre le forze di polizia al fine di scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica, disperdevano i tunisini, liberando completamente l'area. Gli immigrati, scortati dalle forze di polizia, rientravano al centro di Contrada Imbriacola. Nell'occasione sono rimasti contusi una decina di tunisini ed altrettanti appartenenti alle forze dell'ordine. Aggiungo inoltre che il 22 settembre il commissario delegato per l'emergenza ha comunicato di aver pubblicato un bando di gara per l'affidamento dei servizi di rimozione, trasporto, demolizione e smaltimento di imbarcazioni e relitti presenti sull'isola. Inoltre, con provvedimento del 24 settembre scorso il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa ha dichiarato il porto di Lampedusa luogo non sicuro per lo sbarco di migranti ai soli fini del soccorso in mare. Sulla questione, il Ministero dell'interno ha anche chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato che, sulla base delle Convenzioni internazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, ha chiarito il concetto di luogo sicuro di sbarco. Questo viene individuato in località in cui le operazioni di soccorso possono ritenersi concluse, dove la vita delle persone soccorse non è ulteriormente minacciata e dove le loro necessità primarie come cibo, riparo ed assistenza medica possono essere reperite. Ai fini che interessano è dunque da ritenersi essenziale che lo sbarco debba avvenire in un luogo in cui i migranti soccorsi in mare possano essere raccolti e possano avere accesso ai loro bisogni primari. Sin qui i fatti. Dall'inizio di quest'anno sono complessivamente sbarcati nelle isole Pelagie 51.596 cittadini extracomunitari, su un totale di sbarchi, su tutto il territorio nazionale, pari a 60.656 immigrati. Le iniziative e le attività che il Ministero dell'interno ha attuato per far fronte alle emergenze si collocano nel solco della tradizione politica italiana in materia di immigrazione, che è tra le più avanzate in Europa ed è in linea con le previsioni del Patto europeo sull'immigrazione e sui diritti d'asilo. Nella gestione del fenomeno dell'immigrazione, il Governo italiano ha sempre messo in primo piano la salvaguardia della vita umana in mare, numerosi sono stati in tal senso gli interventi dei nostri dispositivi navali anche al di fuori della nostra zona SAR laddove non intervenivano i Paesi convenzionalmente competenti. Sul piano interno, di fronte ad un fenomeno di tali proporzioni, è stata pianificata una serie di misure volte a garantire non solo l'accoglienza dei profughi, grazie all'intesa del Governo con le Regioni ed al ruolo svolto dalla Protezione civile, ma anche la sicurezza del territorio e delle frontiere. Il Governo ha adottato una strategia di contenimento e di prevenzione del fenomeno, con il duplice obiettivo di difendere la sicurezza delle frontiere e di salvaguardare la sovranità dello Stato attraverso il controllo del territorio. territorio. Per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina il Governo ha promosso, e continua a ritenere fondamentale, lo sviluppo e la cooperazione con i Paesi di origine e/o di transito degli immigrati illegali. Sono stati stipulati, come è noto, accordi bilaterali con molti di questi Paesi, in particolare Nigeria, Ghana, Niger, Senegal e Gambia. Particolarmente intensi sono i rapporti di collaborazione con la Tunisia, con l'Egitto e con l'Algeria, Paesi da cui tradizionalmente provengono consistenti flussi di immigrati e che si sono impegnati a contenere le partenze, a collaborare in materia di riammissione e rimpatrio e ad eseguire specifici programmi di assistenza tecnica. Per quanto riguarda la Libia, devo ricordare che, dopo i recenti avvenimenti, il Governo italiano e il Consiglio nazionale transitorio libico hanno firmato a Napoli, il 17 giugno 2011, un *memorandum* d'intesa. Il Ministero dell'interno ha assicurato la propria disponibilità a partecipare all'attività di riorganizzazione delle forze di polizia civili della nuova Libia, curando eventualmente l'organizzazione di corsi di formazione per il personale dirigente e per i formatori. Per quanto riguarda la Tunisia, il 12 settembre scorso il ministro Maroni si è recato a Tunisi per incontrare le autorità di quel Paese. Nell'occasione si è preso atto dei risultati positivi finora raggiunti nella collaborazione con l'autorità tunisina a seguito dell'Accordo del 5 aprile ultimo scorso, e si è concordato di intensificare le operazioni di rimpatrio, prevedendo 10 voli a settimana articolati su cinque giorni, con 100 cittadini tunisini rimpatriati al giorno. Il piano straordinario ha la durata di tre settimane. Ho avuto già occasione di sottolineare, nell'immediatezza dell'evento, come gli atti vandalici e le rivolte poste in essere dai cittadini tunisini siano da mettere in stretta correlazione con la loro consapevolezza di essere rimpatriati. Oggi non posso quindi che ribadire quanto detto in quell'occasione, sottolineando una volta di più che gli episodi, nei cui confronti è ferma la condanna, non hanno modificato e non modificano il piano di rimpatrio, che prosegue e non subirà rallentamenti. Sull'isola oggi non sono più presenti cittadini stranieri irregolari; dalla metà di settembre, ovvero da quando si è deciso e concordato di intensificare le operazioni di rimpatrio, a ieri, sono stati rimpatriati a Tunisi 841 extracomunitari clandestini di nazionalità tunisina. Complessivamente, dal 1° gennaio a ieri sono stati effettivamente rimpatriati dal Viminale 16.566 cittadini stranieri. Per completezza di informazione, ricordo che nella mattinata del 27 settembre scorso tutti i minori presenti sull'isola sono stati imbarcati sulla nave Palladio, diretta a Porto Empedocle, per essere trasferiti presso una struttura ricettiva ubicata a Borgetto, in provincia di Palermo. In conclusione, desidero ribadire quanto più volte ricordato in quest'Aula e nelle sedi istituzionali europee: l'emergenza, che da tempo stiamo gestendo, non è solo una questione da affrontare, come stiamo facendo, al massimo delle possibilità a livello nazionale, ma corrisponde ad una crisi geopolitica che coinvolge tutto il Mediterraneo, e quindi tutta l'Europa. Bisogna comprendere ciò se vogliamo un'Europa capace di costituire un unico grande sistema di governo del fenomeno dell'immigrazione. Ritengo sia un dovere di tutti gli Stati membri aiutare i Paesi sottoposti a particolare pressione migratoria, come è l'Italia oggi, non soltanto sotto il profilo di un'equa ripartizione degli oneri ma anche per quanto concerne l'assunzione di responsabilità da parte dei singoli Stati. L'immigrazione rappresenta una sfida europea e richiede pertanto una risposta europea. Infatti, è soltanto una gestione concordata della crisi, nell'ottica della sussidiarietà e della responsabilità da parte di tutti gli Stati, che può incarnare il vero spirito dell'Unione europea. Occorre tuttavia riconoscere, con obiettività e onestà intellettuale, che questa risposta ancora tarda a venire.

Signora Presidente, le comunicazioni del Governo, delle quali diamo atto alla Sottosegretario, rafforzano l'impressione che tutta la questione relativa a questo tipo di immigrazione andrebbe affrontata diversamente. La posizione geografica dell'Italia, e in essa di Lampedusa, e la funzione politica del nostro Paese nel Mediterraneo non possono risolversi in un assurdo arroccamento, del quale i centri di vario tipo e denominazione da un lato e la latitanza internazionale dall'altro lato sono preoccupante espressione. In effetti, mi pare che anche la non encomiabile rappresentazione in corso sulla nomina del nuovo Governatore della Banca d'Italia contribuisca a far capire come l'interesse nazionale non sia propriamente centrale nell'azione dell'attuale Governo. In una mozione approvata dal Senato lo scorso 29 giugno 2011, questo Gruppo aveva delineato la tematica sostanziale ed aveva elencato alcune proposte operative. Ad esse rinvio, data la brevità del tempo a disposizione. Certo, occorre applicare un ragionevole, distinto giudizio sulle più recenti ondate migratorie, dalla prima dei tunisini a seguito della rivolta che li portava in Italia, quasi l'Italia fosse un pontile verso la Francia, alla seconda ondata libica, di cui Gheddafi ha fatto una vera e propria arma da guerra, che ha visto protagoniste le popolazioni subsahariane lasciate sulle coste ed ha registrato centinaia di morti in mare. Da ultimo, una volta bloccato il flusso dei clandestini dalla Libia, con gli atti di violenza a questo collegati, si è tornati al flusso con i tunisini, perché evidentemente l'accordo bilaterale non ha funzionato, stanti le difficoltà economiche di intere fasce di popolazione di quel Paese. Preso atto che le motivazioni delle ondate migratorie sono diverse, anche l'approccio deve essere differente. Adottare un approccio omogeneo al problema è quindi sbagliato. Naturalmente, occorre applicare tutto il necessario rigore nei confronti di ogni e qualsiasi atto di violenza. Questo va, tuttavia, accompagnato da una più rapida ricognizione dell'identità e dello *status* dei migranti già sbarcati in Italia, garantendo priorità e tutele ai richiedenti asilo politico ed ai profughi di guerra e, soprattutto, ai minori. La concessione del permesso temporaneo rappresenta anche una garanzia per meglio gestire la presenza di immigrati in territorio italiano. In tal senso, come ha affermato anche la Sottosegretario, l'Italia dovrà spendersi in sede europea perché sotto questo profilo i partner dell'Unione europea si dimostrino effettivamente solidali, ben oltre le dichiarazioni di principio. Infine, il pensiero torna a Lampedusa ed a quella popolazione così provata. Nella capacità di sopportare oltre ogni limite, nella capacità di essere comunque accoglienti, i lampedusani hanno espresso una virtù nazionale, quella della solidarietà. Per riconoscerla, la recente proposta di candidatura del film di Crialese all'Oscar vale forse di più dell'improvvisato annuncio di una ipotetica candidatura di quell'isola al premio Nobel.

succedono fatti come quelli accaduti a Lampedusa con ciclico ritmo, irregolare, ma avvengono; ogni volta qualcheduno dei parlamentari chiede che il Governo si presenti a rispondere su questo, e di solito riceviamo delle risposte, non tutte garbate come la sua - ma da quando lei è Sottosegretario le risposte sono di questo tono - che illustrano da vicino il fatto conchiuso, in sé: la Polizia ha fatto questo, i cittadini quell'altro, il questore si è adoperato, le navi sono arrivate, gli aerei sono stati spostati, non si può fare a meno di notare come questa sorta di restringimento ad un tema estremamente limitato come il fatto in sé generi un senso di impotenza interpretativa, perché si perde di vista completamente il contesto, anche quello ravvicinato, in cui tutte queste cose accadono.

non è tutta rappresentata dalle frasi che ho sentito. Ho qui una lettera di un cittadino di Lampedusa - che sarei contento di farle avere - che testimonia come anche lì ci sia chi vede con spirito critico quello che è accaduto e non lesina critiche alla gestione del molto discusso sindaco di quel Comune. il contesto della gestione e dell'impostazione. Noi viviamo sotto la spada di Damocle di una politica che è all'origine

Il timore è che quando siamo collocati in una situazione di questo tipo sia difficilissimo evitare fenomeni come quelli che lei ci ha descritto,

In realtà però l'Italia è la sponda di questo processo di immigrazione e ha di fatto su di sé il carico di affrontare con maggior chiarezza questa faccenda. Non è possibile semplicemente proteggersi dietro l'operato di due commissari di Polizia e del Parlamento europeo, che a un certo punto dovrà garantire una palingenesi di tutto questo fenomeno;

è un errore d'impostazione basilare, dovrebbe prendere atto che il fenomeno dell'immigrazione va affrontato con altri mezzi, e l'opposizione su questo - non ho più il tempo di dirlo - ha già avanzato proposte profondamente diverse

Voglio ringraziare in particolar modo le forze dell'ordine, a cominciare dal prefetto e dal questore e, in particolare, un Corpo che viene sempre trascurato nei ringraziamenti, quello dei Vigili del fuoco, che hanno operato in maniera egregia. Ho ascoltato con attenzione la sua relazione, e le dico subito che nell'emergenza il Governo si è comportato e

nelle navi per giorni. Per il resto mi sembra che non si potesse fare altro. Qualche tempo fa, parlando con il vescovo italiano a Tunisi, tentavo di avere da lui qualche indicazione sul fatto che l'emergenza in Tunisia fosse finita, perché la rivolta e la contestazione a quel Governo erano ormai superate. Ma la risposta del vescovo fu precisa:

Se questo è vero, non possiamo rimanere legati all'emergenza, che pure - glielo dico ancora una volta - è stata gestita bene, ma bisogna pensare a una pianificazione.

Benissimo sottolineare che l'Europa è colpevolmente assente nella gestione è doveroso che i nostri Ministri si facciano sentire in Europa; però anche su questo punto ho poche speranze che un giorno l'Europa possa venirci in qualche modo incontro. Questo è allora un problema che dobbiamo pianificare noi, e tale pianificazione francamente lascia a desiderare. Raggruppando tutta questa gente in un'isola, quanto potrà durare la pazienza degli isolani? Lampedusa non è più un porto sicuro, ma la domanda è: ma coloro che sono in mare intorno a Lampedusa che devono fare, dove vanno a parare?

ringraziare tutti i colleghi, perché evidentemente questo argomento interessa solo pochi, visto che l'Aula è completamente vuota. L'isola di Lampedusa sta vivendo ormai da troppo tempo un periodo di continui sbarchi di migranti irregolari, che la danneggiano e mettono a rischio l'incolumità di noi abitanti. Sono assolutamente d'accordo con l'iniziativa del ministro Maroni per quanto riguarda la politica di espulsione e gli accordi assunti, in particolar modo dopo quanto è avvenuto sull'isola una settimana fa. queste persone hanno dimostrato di essere pericolose per Lampedusa, ma sarebbe anche un rischio far sì che si disperdano incontrollate per il nostro Paese. Cari colleghi, dovete sapere che l'episodio

Per quanto riguarda l'esposto presentato a Palermo a proposito di quelli che vengono definiti *lager* galleggianti, il Ministro ha ben operato,

(come è successo a due marinai, che da una settimana non portano un pezzo di pane a casa perché hanno rubato loro il peschereccio). Bisognerebbe infatti preoccuparsi di denunciare, piuttosto, tutte le questioni che affliggono il Mezzogiorno, prima fra tutte quella della disoccupazione che, come evidenziato dai dati ISTAT, fa registrare nel Sud del nostro Paese il tasso più alto di disoccupati. È per tale ragione che le già poche risorse esistenti devono essere utilizzate per affrontare innanzitutto i problemi che gravano sulla nostra di popolazione. Dal momento che questa emergenza è gestita unicamente da noi senza aiuti da parte del resto d'Europa, io non tollero critiche sulla gestione di tale fenomeno, ma chiedo solamente al Ministro di continuare così, e lo faccio perché questo è il volere della maggior parte degli italiani e soprattutto dei lampedusani che non possono più sopportare questi abusi. Sì, perché di abusi voi non potete capire cosa significa affrontare questi delinquenti che minacciano di far esplodere un distributore di benzina con una bombola di gas aperta. Tutto questo deve finire: dobbiamo iniziare a far sentire la nostra voce per evitare che per la loro salvezza venga sacrificata la libertà e la salute, non solo dei lampedusani, ma di tutto il nostro Paese.

Si spera che Lampedusa non continui ad essere quell'Isola del Diavolo della Caienna che è stata per nove mesi, ma in futuro che cosa si farà? Quali sono le idee politiche del Governo? Su questo punto vi è un'enorme carenza.

sufficiente. Ricordiamo che il Sud della Tunisia è stato gravemente disastrato dalla guerra con la Libia, dalle centinaia di migliaia di profughi transitati dal Sud, dalle centinaia dalle centinaia di migliaia di tunisini rimpatriati, dalla fine di tutto il traffico transfrontaliero che dava sostegno alle popolazioni locali, dalla chiusura delle attività turistiche. La Tunisia è un Paese sull'orlo del baratro economico: noi sappiamo che è così. Il nostro Paese deve in qualche modo farsi carico di interventi più a largo raggio, che non siano quelli delle motovedette e dei pattugliatori. Questo è un grossissimo problema, che va affrontato. Non ho sentito una parola della sottosegretario Viale su questi temi, che rilevano enormemente sul futuro dei nostri rapporti con la Tunisia. Certo, noi vorremmo avere la Svezia invece della Tunisia dall'altra parte del Mediterraneo, ma la geografia ha voluto altrimenti, e credo che di questo bisogna farsi carico. Per quanto riguarda l'Europa, è ricominciato il piagnisteo, la lamentazione dell'assenza dell'Europa: ma di quale Europa parliamo? Quale credibilità abbiamo noi in Europa se per mesi e mesi non abbiamo avuto un Ministro per le politiche comunitarie?

chi va a rappresentarci in Europa? Quale credibilità ha il nostro Presidente del Consiglio e quale credibilità ha oggi il nostro Paese, che è stato scavalcato su tutte le questioni relative alla Libia e all'intervento in Libia, è messo da parte, e anche umiliato, in sede internazionale? Quindi, l'Europa. Dov'è l'Europa? Cosa facciamo noi per l'Europa? Noi imploriamo la condivisione degli oneri chiedendo

e anche ricordando alla senatrice Maraventano che sul Corriere della sera del 22 settembre è riportata una sua dichiarazione nella quale chiedeva al ministro Maroni l'allontanamento dall'isola dell'«ONU e delle organizzazioni che lavorano per gli immigrati: se ne devono andare,

ampia ed articolata come è stato riconosciuto da tutti, lei ha messo in evidenza tutti i fattori sensibili del fenomeno dei flussi migratori, dalla latitanza dell'Unione Europea. Al riguardo mi permetto di dissentire dalle parole del senatore Livi Bacci perché è apparso a tutti evidente come l'Unione Europea abbia abbandonato l'Italia nell'affrontare questa drammatica drammatica emergenza. Non saranno i numeri differenti tra noi, la Germania e la Francia a consolarci. Per noi questo è un problema grave e serio e registriamo che l'Unione Europea, oltre alle belle parole, non riesce a dire altro

emerge in tutta la sua importanza il carico insopportabile per la povera terra di Lampedusa, che passa però per l'encomiabile capacità di accoglienza della gente italiana, la gente di Lampedusa.

coloro che più di altri e di ogni altra Forza armata e di polizia riuniscono le doti di controllo del territorio alla grande umanità, che è la cifra di questa vicenda, come ci ha dimostrato la gente di Lampedusa. A quella straordinaria popolazione abbiamo l'obbligo di garantire maggiore sicurezza: questo ha messo in evidenza la senatrice Maraventano,

nella fermezza, soprattutto civiltà. Sono certa che questo è il segno attraverso cui passa la gran parte della nostra politica sui flussi migratori e di quella così bene rappresentata da lei, signora Sottosegretario, e dal ministro Maroni.

anche su richiesta del presidente Dini, illustro la relazione al posto del collega Marcenaro, che ha avuto un problema e oggi non può essere presente. Il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo che emenda la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa nel 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e quelli appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il Protocollo risponde alla finalità di armonizzare i contenuti della Convenzione del 1988 al nuovo modello dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni nel campo della fiscalità. Lo strumento dell'Accordo multilaterale tende a fornire alle amministrazioni fiscali degli Stati aderenti strumenti di maggiore efficacia per la lotta all'evasione fiscale a livello nazionale ed internazionale, mediante un costante flusso informativo e alla reciproca assistenza nel recupero dei crediti di natura tributaria. Dall'Accordo non deriveranno oneri finanziari. Inoltre, si prevede che dall'entrata in vigore del Protocollo derivino vantaggi per l'erario, connessi ad un maggiore introito fiscale, stanti le finalità del protocollo di incrementare il contrasto all'evasione fiscale e di sostenere la cooperazione tributaria multilaterale. La tematica del contrasto all'evasione fiscale è direttamente connessa a quella della disciplina del segreto bancario. A tale ultimo proposito, la via privilegiata di regolamentazione è quella dell'Accordo bilaterale. Credo sia superfluo mettere in evidenza l'importanza strategica di questo Accordo e, più in generale, di tutte le politiche sia multilaterali, sia bilaterali per la cooperazione in materia fiscale, anche per combattere e contrastare i cosiddetti paradisi fiscali e quindi i trattamenti di favore inaccettabili nei confronti del fenomeno dell'evasione o addirittura della frode fiscale. In questa direzione, mi piace ricordare l'impegno della Commissione esteri del Senato per rimettere in moto il negoziato bilaterale con la Svizzera, che sta dando segni incoraggianti di ripresa. la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Nell'altro ramo del Parlamento è stato accolto un nostro ordine del giorno a firma del collega Di Stanislao, nel quale, approfittando del passaggio in Aula di un provvedimento come questo, il Governo si è fatto impegnare ad azioni concrete anti-evasione anche e soprattutto all'interno dell'ordinamento italiano dove, ad opinione di Italia dei Valori, occorre urgentemente porre rimedio. Inoltre, questo Protocollo consente di aprire la Convenzione all'adesione di Stati non non membri dell'OCSE né componenti del Consiglio d'Europa, prevedendo un'apposita procedura in questo senso. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009

e quello sudafricano iniziata ormai da molto tempo. Il Sud Africa è un importante partner commerciale per l'Europa e per l'Italia, considerato che è incluso negli ormai famosi BRICS, i Paesi emergenti che oggi guidano la classifica mondiale della crescita economica e dello sviluppo economica e dello sviluppo (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa). Un Accordo di grande rilevanza tra Unione europea e Sud Africa riguardante gli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, che costituisce la cornice principale dei rapporti trai due Paesi, è stato siglato già l'11 ottobre 1999 e l'Italia lo ha recepito nel 2003. La ratifica che prendiamo in esame oggi con l'approvazione dell'Atto Senato n. 2859, attraverso la modifica di un Accordo siglato l'11 settembre 2009, permette di allineare il precedente Accordo dell'ottobre 1999 all'evoluzione del quadro giuridico internazionale, che ha riguardato *in primis* la revisione della cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico, nonché l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale e la lotta contro il terrorismo internazionale avviata dal 2001. Il nuovo Accordo bilaterale aggiornato implementa dunque il precedente del 1999 tenendo conto di queste importanti innovazioni. In maggiore dettaglio, il provvedimento sottoposto oggi a ratifica aggiunge alcune parti di sostanziale rilevanza: anzitutto, il tema della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, per cui viene riconosciuta la vitale importanza del sistema dei Trattati multilaterali sul

pertanto, il rinnovato impegno ad aderire ai predetti Trattati recependo e rispettando gli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, oltre che quello di creare e mantenere un sistema efficace di controlli all'esportazione e al transito di armi di distruzione di distruzione di massa, ponendo particolare attenzione all'impiego finale delle cosiddette tecnologie di duplice uso con sanzioni efficaci nei casi di violazione. In secondo luogo, un'altra delle particolarità della ratifica in esame è la lotta al terrorismo, che viene giudicato criminale, ingiustificato e condannato con fermezza in tutti gli atti, metodi e pratiche, indipendentemente da chi e dove siano commessi. Il nuovo Accordo ribadisce l'importanza della strategia globale antiterrorismo dell'ONU, la volontà di realizzarne gli obiettivi e l'impegno al raggiungimento di un accordo sulla Convenzione generale sul terrorismo internazionale. Sul piano più concreto del contrasto alle attività terroristiche, l'Accordo contiene un impegno alla cooperazione, in particolare nel quadro della risoluzione n. 1373 del 2001 del Consiglio di Sicurezza nelle Nazioni Unite, allo scambio di informazioni e alla reciproca assistenza amministrativa e tecnica nella lotta al riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite e al finanziamento del terrorismo. Tutto ciò attraverso un sistema fatto di adeguate disposizioni, norme e meccanismi di controllo. L'Accordo riconosce però anche l'importanza di combattere combattere alle radici le cause di diffusione del terrorismo e impegna in questo senso le parti allo sviluppo e all'attuazione dei programmi di azione globali volti all'eliminazione delle predette cause. L'Accordo recepisce inoltre il concetto che la lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani non sono obiettivi in contrasto tra di loro e che la prima va condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali e delle leggi dello Stato di diritto. Analoghe norme riguardano il contrasto alla produzione, al traffico e allo stoccaggio delle armi leggere e di piccolo calibro, nonché il contrasto al crimine organizzato, alla corruzione e all'impiego dei mercenari nei conflitti armati. In terzo luogo, si riafferma il sostegno alle attività della Corte penale internazionale quale importante strumento per garantire il rispetto delle decisioni degli organi di giustizia internazionali e porre fine alle impunità. infine gli impegni alla cooperazione in materia di immigrazione, che riguardano il rispetto dei diritti umani dei migranti (di cui oggi abbiamo parlato), la garanzia di non discriminazione, la tutela contro il razzismo e la xenofobia; riguardano altresì la messa in campo di strategie per la riduzione della povertà e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei migranti, ma anche la prevenzione dell'immigrazione clandestina e delle altre attività illecite connesse ad essa, condotte dalle reti di trafficanti, quali il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Concernono dunque la reciproca assistenza tecnica e la condivisione delle *best practice* nella formazione e nello sviluppo delle capacità di controllo delle frontiere. L'Accordo impegna le parti ad assicurare reciprocamente ai cittadini dei Paesi appartenenti all'Unione europea residenti in Sud Africa e viceversa parità di trattamento nel campo del lavoro, in termini di condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamenti. La nuova intesa non concerne approfonditamente la materia degli scambi commerciali. Quest'ultima, infatti, troverà ampio spazio nell'ambito di un più ampio Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e tutti i Paesi dell'Africa australe rappresentati dalla *Southern African Development Community*. Tuttavia, importanti clausole riguardano la liberalizzazione del commercio in alcuni specifici settori, nonché impegni di cooperazione nel campo delle telecomunicazioni, delle politiche energetiche e del trasporto aereo, ferroviario e marittimo (soprattutto in tema di sicurezza dei trasporti) e dei relativi sistemi di navigazione satellitare.

dell'Accordo è previsto esplicitamente che imprese private dei due Stati possano produrre e scambiare non meglio

un salto di qualità che l'Europa mi sembra stia cercando di fare dal punto di vista della politica estera. Parafrasando Galileo, si potrebbe dire che l'Europa, anche quando sembra ferma, «Eppur si muove!».

il provvedimento reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e lo Stato del Qatar, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, il quale riveste una particolare rilevanza dal punto di vista politico nell'attuale congiuntura diplomatica internazionale. La cooperazione in materia di difesa con il Qatar si inserisce, infatti, in un contesto che vede tale Stato particolarmente impegnato in numerosi scenari di crisi. Basta ricordare l'importante funzione che da ultimo le Forze armate qatariane stanno svolgendo nel quadro della missione militare in Libia. Le forze aeree hanno partecipato sin dall'inizio all'appoggio delle operazioni del Comitato nazionale transitorio libico per la presa del controllo della Cirenaica e della Tripolitania. Nonostante le ridotte dimensioni dello Stato del Qatar, l'Accordo bilaterale in discussione pone le basi per una proficua collaborazione nell'importante materia degli armamenti e della difesa. I contenuti dell'Accordo riguardano, infatti, le materie degli appalti nel settore militare, dell'importazione, esportazione e trasporto di armi, dell'applicazione dei Trattati internazionali sulla sicurezza e la difesa e della partecipazione ad operazioni umanitarie e a missioni di pace. In concreto, la cooperazione si articolerà in periodiche riunioni dei rispettivi vertici politici e militari e in attività congiunte di formazione ed esercitazione. Lo scambio di materiale bellico (armi e munizioni) potrà avvenire anche direttamente tra i due Stati ovvero tra aziende private previa autorizzazione governativa. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca una copertura finanziaria pari a euro 12.245 annui, connessi agli oneri per lo svolgimento delle consultazioni, da svolgere alternativamente a Doha o a Roma,

non c'è un problema di rifinanziamento nel senso che è stato cancellato l'intervento.

c'è una coincidenza di fondo, escludendo il problema citato prima rispetto al rifinanziamento e all'applicazione dell'Accordo sulle mine.

proprio nel testo dell'Accordo è previsto esplicitamente che imprese private dei due Stati possano produrre e scambiare non meglio identificate e specificate mine. Come giustamente ha ricordato il rappresentante del Governo, abbiamo trattato questo argomento e abbiamo anche votato,

mine. L'impegno preciso, già assunto dal Governo alla Camera dei deputati proprio su richiesta dell'Italia dei Valori, di valutare l'opportunità di un maggior controllo sulle relazioni che intercorrono tra gli Stati e le imprese private in materia di scambio di armamenti credo debba

a questo Atto del Senato, relativo alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Qatar sulla cooperazione nella difesa. L'Italia dei Valori

questo Atto. Sia chiaro che con il Qatar abbiamo da poco ratificato anche altri accordi, quali quello sulle doppie imposizioni, quello sulla cooperazione culturale e, al pari di quanto già fatto con altri Paesi, oggi anche nel campo della difesa. Sia ancora più chiaro, colleghi, che riteniamo strategica la *partnership* con questo Paese, importante attore, seppur non del tutto democratico, dell'area mediorientale. Ricordo che lì ha sede Al Jazeera. Ricordo che il Qatar è stato il primo Stato arabo ad avere garantito il proprio sostegno in Libia al fianco della NATO. Senza ripetere quanto già contenuto nella relazione del relatore, ribadiamo la non contrarietà allo sviluppo della cooperazione bilaterale, con lo scopo di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Riteniamo che la sottoscrizione di accordi bilaterali come questo rappresenti anche una parallela azione stabilizzatrice. L'impegno già assunto dal Governo alla Camera dei deputati, su richiesta dell'Italia dei Valori, a valutare l'opportunità di un maggior controllo sulle relazioni che intercorrono tra gli Stati e le imprese private in materia di scambio di armamenti, come ho già detto, è da noi ritenuto insufficiente. È per questo che abbiamo presentato l'ordine del giorno G101 (poi trasformato in una raccomandazione), con il quale si impegnava il Governo a modificare puntualmente l'Accordo in questione. Per tutti questi motivi, l'Italia dei Valori voterà

Crosetto - che contengano l'esplicita autorizzazione a produrre e a scambiare mine, con Paesi neppure democratici. Il tutto, in un quadro che vede, dal 2001 ad oggi, una riduzione pressoché totale dei fondi per lo sminamento umanitario. Dall'entrata in vigore della legge, approvata dal Governo Amato nel 2001, le dotazioni del fondo, per alcuni mesi addirittura azzerate, sono scese e sono ora ad un quinto di quanto destinavamo, appunto, nel 2001. Facendo appello alla Presidenza del Senato affinché per il futuro, sul sito Internet dell'Istituzione, sia sempre possibile visionare anche i testi degli Accordi (ribattuti o fotografati: non è importante),

Signora Presidente, noi voteremo a favore di questa ratifica perché crediamo nel valore della cooperazione anche sul terreno militare, in particolare con un Paese amico com'è il Qatar. Basti pensare al comune impegno che ha visto l'Italia a fianco del Qatar nell'attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite sulla questione della Libia.

Possiamo dedurre da una serie di elementi e di indizi sul campo che il Qatar in questo momento sembra appoggiare alcune forze in Libia che sostengono

in Qatar, e questo è uno strumento di straordinaria importanza per l'evoluzione, o l'involuzione, del mondo arabo-islamico). Allo stesso tempo, accanto a questa mano tesa ci vogliono elementi di cautela e di prudenza. È per questo che abbiamo proposto l'ordine l'ordine del giorno G100, che il Governo ha accolto (e di questo ringrazio il sottosegretario Scotti): proprio perché, trattandosi di una materia così sensibile come quella della cooperazione militare, in un contesto non privo di preoccupazioni, in particolare sul versante dei dei diritti umani, credo sia giusto da parte dell'Italia far sapere ai nostri amici del Qatar che la nostra cooperazione e la collaborazione che offriamo, in particolare in un settore così sensibile come quello militare, non è senza condizioni. La condizione fondamentale è che la forza del Qatar - quella economica che è molto imponente, quella culturale che è molto forte, con Al Jazeera, e anche quella militare, che anche con il nostro concorso va a rafforzarsi - sia messa al servizio della democrazia e dei diritti umani e non dei loro nemici. Signora Presidente, dopo la precisa, puntuale e brillante relazione del collega Amoruso, il mio Gruppo voterà favorevolmente all'Atto Senato n. 2857.

una nuova finestra") ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,

Signora Presidente, il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra Unione europea e Indonesia, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, riveste una particolare importanza, poiché si tratta dell'istituzione di un Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione. il primo Accordo di questo tipo che viene sottoscritto dall'Unione europea con uno Stato dell'area dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni dell'Asia sudorientale) e costituirà il riferimento per eventuali futuri accordi con altri Paesi della regione. L'Accordo pone le basi per un nuovo quadro giuridico di riferimento per la cooperazione tra Europa ed Indonesia, la quale viene considerata un *partner* strategico tanto dal punto di vista politico quanto da quello economico, ove si considerino i tradizionali legami di quell'area con la Cina e con gli Stati Uniti. A livello contenutistico, l'Accordo individua una serie di principi generali che si rifanno alla democrazia e al rispetto dei diritti umani fondamentali, nonché ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile e ad affrontare le sfide del cambiamento climatico; specifica menzione è fatta ai principi del buon governo e dello Stato di diritto. Le finalità della cooperazione sono quelle di rafforzare le relazioni bilaterali e a mantenere un dialogo globale, nelle sedi e organizzazioni sovranazionali, nonché quelle di perseguire lo sviluppo degli scambi e degli investimenti. L'Accordo si articola in cinquanta disposizioni suddivise in sette titoli che riguardano specificamente quattro aree di cooperazione: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia. Il disegno di legge reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, poiché dall'Accordo non derivano ulteriori oneri finanziari a carico degli Stati membri rispetto a quelli che verranno assolti a livello di Unione europea. Come avevo detto prima a proposito del Sud Africa, anche questo Accordo quadro è un segno importante della politica estera che l'Unione europea sta cominciando a costruire a livello internazionale, in particolare con queste nuove potenze emergenti. L'Indonesia è il più grande Paese islamico del mondo dal punto di vista della popolazione ed è una vera e propria potenza economica emergente. Quindi credo che sia assolutamente assolutamente importante e strategico questo Accordo con l'Unione europea nel suo insieme. Per tutte queste ragioni, la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Signora Presidente, il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica, già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, dell'Accordo concluso tra Italia e Giordania nel novembre 2007, volto alla prestazione di assistenza e cooperazione reciproca ai fini del rispetto della legislazione doganale e alla realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi. Giova ricordare il consistente interscambio commerciale che esiste tra Italia e Giordania, nonché il ruolo strategico che tale Stato svolge nello scenario regionale. Quanto ai contenuti dell'Accordo, la collaborazione nel contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti. Specifiche disposizioni sono dedicate all'individuazione delle autorità competenti, all'applicazione dei nuovi obblighi, allo scambio informativo e alle attività di prevenzione del contrabbando e del traffico illecito di merci e di beni artistici. Viene regolata l'assistenza a livello informativo e di individuazione e punizione dei responsabili di infrazioni. Il disegno di legge reca una copertura finanziaria pari a euro 11.325 annui a decorrere dal 2011. La Commissione propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea

riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010***

di partenariato nell'ambito dei rapporti tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (i cosiddetti Paesi ACP). L'atto di base è rappresentato dall'Accordo di Cotonou del 2000, il quale, essendo soggetto a revisione quinquennale, è stato aggiornato una prima volta a Lussemburgo nel 2005 e viene ora nuovamente modificato. L'Accordo tende in particolare all'adattamento del quadro normativo relativo ai rapporti fra l'Unione europea e i Paesi cosiddetti ACP rispetto ai mutamenti che si sono verificati nelle relazioni internazionali. Le modifiche introdotte interessano numerose disposizioni del testo normativo e si ispirano a taluni importanti principi di fondo, tra i quali assume un rilievo decisivo quello per cui le politiche di cooperazione allo sviluppo poste in essere dall'Unione europea siano strettamente connesse al rispetto di principi fondamentali quali le libertà politiche e la tutela dei diritti umani. dell'Accordo di Cotonou è stato modificato onde permettere l'adesione del Sud Africa, che non era tra i firmatari dell'originario accordo del 2000. non è prevista una clausola di copertura finanziaria poiché il finanziamento avverrà a valere sul X Fondo europeo di sviluppo, cui l'Italia già contribuisce con un ammontare complessivo di 2.916 milioni di euro. Non si produrranno pertanto ulteriori oneri di finanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.